link apre una nuova finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Senatore Marton, possiamo sensibilizzare il Governo in questo senso e spero che i suoi rappresentanti qui presenti

è stato operato al comma 3 dell'articolo 1, in cui vengono specificate nel dettaglio le risoluzioni delle Nazioni Unite in tema di donne, pace e sicurezza, Grazie accogliendo una sollecitazione proveniente anche dai Gruppi dell'opposizione (e in particolare dal Movimento 5 Stelle), avevamo ritenuto opportuno non enumerare in maniera specifica le diverse risoluzioni delle Nazioni Unite alle quali fare riferimento, per consentire poi implicitamente di acquisirle man mano che eventualmente fossero intervenute. Alla Camera si è invece ritenuto di enumerare in maniera specifica nuovamente le risoluzioni e, dunque, è stato adottato il relativo emendamento con il consenso in quella sede di tutti i Gruppi, salvo quello del Movimento 5 Stelle, che si è astenuto sul voto dell'articolo così modificato. L'altra modifica intervenuta alla Camera alla Camera sottrae al Governo la discrezionalità in relazione all'applicazione del codice penale militare di guerra. Nel provvedimento Nel provvedimento che avevamo approvato al Senato noi avevamo previsto una sostanziale discrezionalità, che invece alla Camera viene vincolata all'adozione di un apposito disegno di legge.

le modifiche intervenute alla Camera e sono queste tre le uniche parti del provvedimento sulle quali il Senato può ulteriormente intervenire. Ovviamente il nostro auspicio, che credo di condividere con il collega Casini, è che l'*iter* del provvedimento si concluda con

la necessità di adottare decreti-legge periodici, che garantisce la copertura delle nostre donne e dei nostri uomini in missione e che definisce in maniera compiuta il rapporto esistente tra i diversi livelli istituzionali in tutta la materia. Inoltre, per l'ennesima volta insisto nel sottolineare l'importanza che sul provvedimento in esame si registri un consenso largo del Parlamento. Ricordo che in Commissione, pur in presenza di articolate votazioni sui singoli emendamenti, si è tenuto un atteggiamento estremamente costruttivo parte delle forze di opposizione. E c'è stato anche un contributo, che è stato preso in seria considerazione - ovviamente nella precedente lettura, quando avevamo margini di modifica

importante, dà lustro al nostro Parlamento e soprattutto ci mette meglio nelle condizioni di assolvere alle nostre funzioni sul piano internazionale,

uno dei più grandi motivi di orgoglio del nostro Paese. *(CoR)*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, la sobrietà e il tono asciutto, per non dire dimesso, della relazione dei colleghi Latorre e Casini non deve togliere importanza

da quel muro che è sembrato insormontabile per quasi mezzo secolo: l'articolo 11 della Costituzione, la questione della pace. Grazie allo strumento di cui il Parlamento - mi auguro - vorrà dotarsi, noi superiamo - vorrà dotarsi, noi superiamo tale muro e dotiamo la nostra politica internazionale del massimo strumento di controllo da parte del Parlamento e di rapidità di decisione da parte dell'Esecutivo. dell'Esecutivo. La nostra politica estera, ormai già da molti anni, ha un suo momento significativo, forse decisivo, nella presenza delle nostre missioni internazionali. Non dico che la nostra politica estera si incentri e si riduca esclusivamente alle missioni internazionali, ma è chiaro che quei cittadini italiani in divisa, che ci rappresentano sul terreno delle organizzazioni internazionali o semplicemente nell'attuazione dei principi di diritto internazionale, sono la nostra politica estera. Ad essi non deve mai mancare il più largo e convinto sostegno del Parlamento, a prescindere da maggioranza e opposizione in politica interna. Riprendo dal collega Latorre due considerazioni, la prima in materia codicistica. Tutto sommato è meglio così: è meglio un eccesso di prudenza e di lentezza in materia di codice, rimettendoci sull'applicabilità sull'applicabilità del codice al disegno di legge del Governo. In secondo luogo, è stato più che opportuno che da parte del Parlamento si sanasse quella ferita di rappresentatività in seno a un organismo parlamentare come il Copasir, che precludeva

un provvedimento organico - come è già stato detto - che sostanzialmente supera il famoso rito dei decreti-legge che arrivano sempre tardivamente e che - a nostro

allertare il Consiglio supremo della difesa; dopodiché saranno le Camere a stabilire l'area geografica, gli obiettivi, la composizione delle forze, il nostro personale, la durata e le risorse che, alla fine, troveranno copertura in legge di stabilità.

da comunicare immediatamente alle Camere. Le Commissioni competenti dovrebbero dare immediatamente l'assenso o viceversa non consentirlo.

giustamente, perché - a nostro avviso - qualora la missione militare internazionale in Afghanistan dovesse cessare, probabilmente quei territori verrebbero rapidamente riconquistati dal controllo di fondamentalisti islamici. Con tutte le connessioni internazionali, lo Stato islamico - che, come abbiamo visto, ha fatto sortite in Libia - non avrebbe difficoltà, al di là delle distanze materiali, avere una consonanza ideologica e nel fanatismo con gruppi che dovessero riconquistare quei territori. È ovvio che la prosecuzione di quella missione, come è emerso nei recenti vertici internazionali della NATO, dovrà trovare nel Parlamento una discussione

parlando di missioni internazionali, a trasportare migliaia di clandestini in Italia. Non scatta però la terza fase, di cui tanto si parla - ovvero la lotta agli scafisti e ai trafficanti in Libia, con la collaborazione del Governo libico - perché le condizioni di agibilità del Governo libico sono scarse.

che il trascorrere del tempo non induce il Governo a una riflessione critica e a una sospensione della missione. Aggiungo, in conclusione, che anche il recente vertice della NATO a Varsavia ha deciso di mandare altre navi a sostegno dell'operazione

il numero delle navi, non essendoci garanzia della terza fase per combattere gli scafisti, è un modo per aiutare una transumanza scomposta e inopportuna, i cui numeri vengono quantificati come

obbliga a una riflessione e a una considerazione sulle criticità, ma anche sulle lungaggini che spesso si hanno su temi così delicati, su cui dovremmo invece essere molto più tempestivi. È chiaro che,

hanno favorito discussioni ampie e partecipate nelle Commissioni di merito. Lo spirito testimoniato è stato costruttivo e collaborativo,

abbiamo dichiarato sempre il nostro voto favorevole, considerata l'importanza della partecipazione dell'Italia a tutto questo e il ruolo che le nostre truppe e i nostri civili impegnati svolgono in ogni teatro dopo le risoluzioni dell'ONU o della NATO. Si tratta di un ruolo importante e determinante, per la capacità dei nostri militari e dei nostri civili anche in termini di umanità, che non si riscontra certamente in altri Paesi. dato altrettanto importante è il fatto che questo provvedimento nasce da una discussione aperta e continua in Parlamento, il che è un buon viatico per far sì che molte cose nascano in Parlamento e non provengano dal Governo. Finalmente abbiamo dato una cornice e una certezza ai nostri militari, che sanno adesso perché agiscono e come agiscono, con regole chiare e con i codici militari di guerra ben delineati. Certamente andrebbe rivisto il trattamento economico, trattandosi di gente che rischia

è accaduto altre volte, un qualsiasi rappresentante del Ministero degli affari esteri. Come fanno le altre Nazioni in queste missioni, credo che la presenza militare debba essere accompagnata da un'azione di politica estera chiara in questi Paesi, per far sì che l'Italia abbia un ruolo determinante e importante, considerato il contributo che offre in termini di uomini, di mezzi, di civili e spesso anche di vite umane. Questo è quello che auspichiamo. Ci auguriamo di poter svolgere un dibattito su

anche noi ci richiamiamo alle dichiarazioni fatte precedentemente in discussione generale. Daremo benevolo assenso a questo provvedimento, che ha visto sostanzialmente anche il contributo della Lega Nord. Rimarchiamo che esiste un'area grigia, dove non è certo quale sia il potere delle Commissioni nel momento in cui divergano rispetto alla volontà del Governo.

che maggiormente garantisce operatività e protezione dai rischi cui inevitabilmente sono sottoposti i nostri militari. Fatte queste osservazioni, che andavano pur dette, anche da parte della Lega Nord ci sarà un voto favorevole.

Signor Presidente, visto il provvedimento che dobbiamo votare, annuncio il voto favorevole di Area Popolare e consegno il testo del

Signor Presidente, colleghi, sarò breve anch'io per non tediare l'Assemblea. Vorrei stigmatizzare per l'ennesima volta l'atteggiamento che ha mostrato il Governo nell'affrontare questo provvedimento. L'unico motivo reale per cui noi siamo ancora, in quarta lettura, a doverci pronunciare sul provvedimento in esame è il fatto che vi sia un accordo tra Forza Italia e il PD per aumentare il numero dei componenti del Copasir. Ci avete fatto lavorare in maniera indegna negli ultimi due giorni; avete fatto calendarizzare il provvedimento in Assemblea prima ancora che in Commissione, dove si è assistito a una farsa. Non si capisce perché alla Camera dei deputati il PD abbia permesso di modificare delle parti che erano fatte bene.

questo non è il modo di lavorare. Ritengo altresì indegno il fatto che si sia utilizzato un disegno di legge per modificare ed aggirare un'altra legge, la n. 124 del 2007, per aumentare di due membri il Comitato parlamentare di controllo per la sicurezza della Repubblica esclusivamente da qui a fine mandato. Voi avete aggirato la legge n. 124 con questo provvedimento esclusivamente per Forza Italia *(Applausi dal Gruppo M5S)*. È una cosa indegna: non si è mai vista una cosa del genere. Vorrei capire cosa vi darà Forza Italia in cambio

sono totalmente in disaccordo sul metodo: bastava semplicemente fare un disegno di legge per modificare la legge n. 124 e sarebbe stato tutto

Signor Presidente, anche noi facciamo una dichiarazione di voto breve, semplicemente per confermare tutte le perplessità

al criterio dell'emergenzialità dei decreti-legge sulle missioni, in realtà l'obiettivo non è stato raggiunto per vari motivi. Quello principale che noi abbiamo rilevato e che abbiamo fatto più volte notare è sicuramente la mancanza e la garanzia di un forte controllo da parte del Parlamento. Ma comprendiamo che anche questo disegno di legge si inserisce molto bene nel disegno più grande di questo Governo, ossia l'accentramento delle funzioni e dei poteri nell'Esecutivo

un ruolo internazionale all'Italia e alla politica estera italiana, per dare una forte copertura e un inquadramento alle nostre vere missioni internazionali, missioni civili e di pace, con pieno riferimento all'articolo 11 della Costituzione, e non invece a missioni con vere e proprie operazioni di bombardamento, come abbiamo visto tra l'altro con il recente decreto-legge missioni approvato poche settimane fa

varie missioni e sull'opportunità di destinazione delle risorse. Invece, anche la scelta di destinare risorse a un Fondo missioni internazionali ancora una volta va a spostare tutta la decisione sulla ripartizione, poi con atti meramente Per noi ancora un volta è stata persa un'occasione in sede internazionale proprio per riconoscere il ruolo del nostro Paese che ripudia la guerra e disciplina l'uso della forza

un lungo percorso legislativo che consentirà finalmente di superare la vetusta disciplina della decretazione d'urgenza in tema di missioni internazionali. Tali missioni rappresentano, come è naturale, un punto qualificante della nostra politica estera, soprattutto in un momento di grave e di elevato rischio per la sicurezza in tutta l'area del Mediterraneo. Nei giorni scorsi in Senato abbiamo espresso il nostro voto favorevole per l'ennesima, forse ultima, conversione di un decreto-legge di rifinanziamento delle missioni. Lo abbiamo fatto come sempre da forza di opposizione responsabile, avendo stima e riconoscenza verso le nostre Forze armate che si distinguono per senso del dovere e alta professionalità, nonostante le continue riduzioni di spesa che il comparto ha sin qui patito. Ora finalmente, dopo parecchi anni, si è forse interrotta la spirale dei tagli al settore difesa che, nel corso degli anni, è sembrato un bancomat cui attingere con più frequenza. Un cambio di rotta comunque ancora limitato se vogliamo che il Paese adempia in maniera adeguata agli innumerevoli impegni internazionali cui è chiamato dovendo nel contempo garantire, attraverso le Forze armate, un'idonea cornice di sicurezza al Paese. Il nostro voto positivo al provvedimento, anche in questa occasione, non mitiga tuttavia l'atteggiamento fortemente critico verso l'operato del Governo in materia di politica estera. Tanto più allorquando aumenta la consapevolezza d'essere esposti, come o più di altri, al rischio del terrorismo sanguinario che continua a mietere vittime innocenti. Un grave e drammatico pericolo agli equilibri mondiali, come non si ricordava dal secondo conflitto. Seguitiamo, pertanto, a ritenere deficitaria la politica estera italiana,

piuttosto che coinvolgerla nella comune e drammatica lotta al terrorismo che incendia il mondo. La stessa cecità nell'avere compreso con estremo ritardo, da parte dell'Alleanza atlantica, che il vero primario pericolo perviene dalla frontiera Sud e non dai confini orientali, come il Parlamento italiano tentava molti mesi fa di far capire al Segretario generale della NATO. Per non parlare dell'avallo alle disastrose primavere arabe, del sostegno in armi e finanziamenti alle forze anti-Assad in Siria, tra le quali anche i gruppi terroristici. Insomma, avrebbero molto da farsi perdonare il presidente Obama, la signora Clinton ed altri "statisti", per così dire, occidentali, manchevoli e lacunosi nelle recenti scelte di politica estera. Sulla stabilizzazione della Libia, pur apprezzando la cautela del Governo italiano, dopo un primo approccio muscolare e bellicista, vorremmo comprendere meglio quali benefici ricaveremo da un Esecutivo libico che in un punto del suo programma politico, presidente Calderoli, ha previsto la *shari'a* quale unica fonte del diritto. Stupisce che nessuno in Italia o in Europa si sia posto il problema del dettaglio della democrazia e dei diritti civili nel prossimo futuro di quel Paese. L'unica certezza, per il momento, è che dalla Libia, pur in presenza di un Governo quasi legittimo, continuano a partire migliaia di persone alla mercé di trafficanti e organizzazioni criminali che lucrano sulla loro disperazione. E tutto ciò anche grazie alle politiche incentivanti dei Governi italiani degli ultimi anni e nonostante le missioni di apparente contrasto varate dall'Unione europea,

ha tradito le ragioni per cui era nata. Con la stessa missione si provvederà nel prossimo futuro ad addestrare guardia costiera e marina libiche, ma quanto tempo trascorrerà per porre un freno all'incontenibile traffico di esseri umani? Quand'è che il neo-*premier* al-Sarraj sarà in grado da solo di controllare le coste libiche? Per quanto tempo ancora sarà consentito, attraverso il traffico di migranti, anche il finanziamento del terrorismo? Siamo certi che il ministro Pinotti non mancherà di porre queste domande al Vice *Premier* libico che nelle prossime ore sarà nel nostro Paese. Consentiteci, perciò, qualche dubbio sulle scelte di politica estera del Governo italiano, nonostante annunciamo il nostro voto favorevole al provvedimento in esame. Abbiamo pianto, Presidente, nei giorni scorsi le ultime vittime italiane nell'attentato di Dacca, ma il Governo italiano in quei giorni, con una scelta infelice ed autolesionistica, ha sospeso la fornitura di pezzi di ricambio degli aerei F-16 all'Egitto, cioè a un Paese amico decisivo in Libia, principale alleato in Nord Africa, del quale siamo anche il secondo *partner* commerciale. Un inutile e dilettantesco gesto ostile, dopo il ritiro dell'ambasciatore, nei confronti di un Paese quotidianamente impegnato nella lotta al terrore che ha mietuto nei giorni scorsi anche vittime italiane. L'unico risultato ottenuto, attraverso un gesto simbolico - dicono dalle parti del PD - è stato quello di innalzare il livello della contrapposizione, che non gioverà né a scoprire i colpevoli dell'omicidio Regeni, né a pretendere nei giusti modi, con fermezza e lungimiranza, la verità, senza imporre a quel Paese una verità precostituita dalle nostre emozioni. Confermiamo comunque il nostro voto favorevole a un importante provvedimento legislativo sul quale Forza Italia si è ben spesa nei due rami del Parlamento, compiaciuti per l'opportuna e tempestiva iniziativa del senatore Latorre che, unitamente ai Presidenti delle due Camere, ha posto rimedio a quell'autentica forzatura per cui un'importante Gruppo di opposizione, quello di Forza Italia, era privato dal partecipare all'organismo parlamentare di controllo sui servizi segreti. Spiace che i colleghi del Movimento 5 Stelle ancora oggi non comprendano quella che era una emergenza democratica. Una questione rilevantissima, divenuta con il tempo non più tollerabile, nel momento in cui il nostro Paese si ritrova impegnato a fronteggiare gravi e pericolose insidie attraverso il lavoro delle nostre Forze armate e quello non secondario dei nostri servizi di sicurezza. Per cui, plaudiamo alla sensibilità del senatore Latorre e al lavoro del Parlamento che, in un delicato frangente geopolitico, è in grado di costruire un clima che offra ai nostri militari impegnati all'estero la gradevole percezione di un Paese unito. *(Applausi

sottolineando però l'importanza di questo momento, perché nella quotidianità del dibattito politico e anche magari rispetto ad alcune deficienze formali che ci sono state anche stamattina nel confronto all'interno delle Commissioni, si rischia di dimenticare che stiamo arrivando in porto con una legge

Stamattina celebriamo qualcosa di molto significativo: le missioni militari sono parte della politica estera e internazionale del nostro Paese; attraverso le missioni agiamo per stabilizzare le situazioni di crisi nell'ambito degli organismi internazionali.

e ci ha lasciato interdetti. Grazie all'intuizione del presidente D'Ascola, in Commissione avevamo raggiunto l'unanimità;

è la fattispecie per evitare che ogni volta che succede una qualsiasi cosa vengano iscritti nel registro degli indagati forze di polizia.

una serie di conseguenze dal punto di vista psicologico, di preoccupazione da parte dei soggetti. Ricordo la tesi secondo la quale dovevamo introdurre un reato di tortura che fosse equilibrato rispetto agli interessi in campo; campo; ho fatto all'inizio un invito a ritirare tutti gli emendamenti e a lasciare solo alcuni degli emendamenti dei relatori. Mi domando allora per quale motivo dobbiamo continuare in un'ottica che improvvisamente si è palesata in Aula, esprimendo parere favorevole ad un emendamento

un qualcosa di diverso e una maggiore possibilità di essere approvato. Quando si parla di un verificabile trauma psichico è è evidente che tutto si regge nel testo votato dalla Commissione e non si può togliere una parte e lasciarne altre. Se doveste fare un'operazione di questo tipo mi porterete a sostenere l'emendamento del collega Gasparri che,

per rappresentare la necessità di una riflessione chiara e precisa. Il Gruppo di Forza Italia, ritirando tutti gli emendamenti

mi permetto d'intervenire soltanto per dar conto delle modificazioni che sono state introdotte e che noi abbiamo ritenuto giusto accertare. Il senatore Caliendo dice la verità e non era possibile pensare altrimenti. Io mi assumo la responsabilità infatti di aver introdotto quel «reiterate». Ciononostante, credo sia manifestazione di umiltà ma anche di disponibilità sentire ragioni contrarie alle proprie iniziali opinioni e aver rivalutato questo contesto normativo. È stato rivalutato proprio alla luce di quello che io già mi ero permesso di dire, ma che

che per la tipicità della condotta sia necessario reiterare, magari in tempi anche diversi, quindi in giorni diversi, le medesime condotte di tortura, determinando ovviamente una tale rarefazione della norma da procurarne la inapplicabilità.

del senatore Caliendo).* Noi abbiamo ritenuto di tutelare le Forze dell'ordine, come è doveroso fare; per questo avevo ritenuto di dire all'esordio che questa è una norma equilibrata, che tiene conto della necessità di tutelare persone destinatarie di condotte violente e offensive, ma anche ovviamente le Forze dell'ordine, per esempio accogliendo quell'emendamento che vuole che intanto la tortura implichi un nucleo iniziale di illiceità. Infatti, il pubblico ufficiale che si mantenga nel perimetro dei poteri e nel rispetto dei doveri connessi alla funzione, ovvero al servizio se si tratta di incaricato di un pubblico servizio, non ha nulla da temere. La locuzione al plurale «violenze e minacce gravi» implica che non potrà mai ritenersi sussistente la tortura se vi è un unico atto. Gli atti devono essere plurimi, quindi non uno solo, ma la reiterazione determinerebbe quel rischio di ritenere quel reato abituale, come i maltrattamenti in famiglia tanto per fare una esemplificazione

quello che avevo già anticipato e quello che per chiarezza, ma anche per manifestazione di umiltà, abbiamo ritenuto di dover precisare. Ripeto che convincersi dell'esattezza delle opinioni contrarie significa seguire i lavori parlamentari e manifestare rispetto nei confronti dell'istituzione parlamentare.

citata, che parla di tortura, in realtà - come ho avuto modo di dire l'altra volta - definisce tortura le minacce gravi che provocano un verificabile trauma psichico, ma le minacce gravi che provocano un trauma psichico sono già tortura.

che lo hanno immobilizzato. Cosa ha detto la sentenza di ieri? Che vi sono state percosse da parte dei carabinieri? Assolutamente no. Che la morte è stata determinata dal delirio da cocaina che, come è noto, quando finisce l'effetto, naturalmente (come hanno scritto tutti i tossicologi) può provocare la morte? Certo, hanno scritto questo. Però hanno dato sette mesi ai carabinieri perché, nel momento in cui - come Preiti davanti a Palazzo Chigi - l'hanno tenuto fermo in terra e gli hanno messo le manette, avrebbero dovuto prevedere

atteggiamenti dolosi. Per cui quei carabinieri che hanno fermato Preiti davanti a Palazzo Chigi, se quel signore che ha sparato al carabiniere e che poi è stato immobilizzato fosse morto, secondo voi dovevano avere l'ergastolo,

da parte delle autorità o da un privato e venga torturata per estorcerle confessioni e farle dire qualcosa che non vuole dire. Certo che il caso Regeni è un caso di tortura. Ma quando leggiamo che qualche procuratore dice che il caso Regeni sarebbe come il caso Cucchi,

E non vanno mica sotto processo, perché dichiarano che l'hanno fermato, ha fatto un movimento di reazione e l'hanno ammazzato. Dio ce ne scampi e liberi da quella concezione delle Forze dell'ordine. Che fanno i carabinieri e i poliziotti italiani quando devono fermare un violento? Lo devono fermare con la forza, rischiando loro, finendo all'ospedale o ammazzati molte volte. E noi introduciamo una norma che automaticamente, in tutti quei casi, consente una denuncia, comprese 'ndrangheta, camorra

se veramente il trauma psichico c'è o no; ma noi automaticamente paralizziamo ogni possibilità di intervento delle Forze dell'ordine. Pregiudizialmente abbiamo già stabilito che, comunque e sempre, nel momento in cui succede un episodio in cui il fermato ha traumi o sfortunatamente, come può capitare, anche per ragioni totalmente estranee (basta leggere le perizie dei tossicologi nel caso di Firenze o in altri casi, purtroppo, di persone che escono dal delirio da cocaina

l'ho già detto: non siamo nel 1925, nella Camera fascista, dove si impediva di parlare; siamo nel Parlamento italiano. chieda la parola e risponda nel merito.

concordato con il Movimento 5 Stelle. Ma vi sembra una cosa seria, quando si parla di ordine pubblico? Voterò con convinzione tutti gli emendamenti che tenteranno di riportare questo testo alla tortura e non a qualcosa di diverso che si vuole inserire per penalizzare e umiliare le Forze dell'ordine.

Senatore Buccarella, ciascun senatore ha il diritto a fare per dieci minuti la propria dichiarazione di voto. *(Applausi dai

nel termine «reiterate». Le argomentazioni del presidente D'Ascola in tema di qualificazione del fatto

Esso deve essere ben dettagliato dal legislatore. La condotta deve essere puntuale e precisa: non la si può lasciare all'interpretazione della giurisprudenza che si formerà su questo testo. Per noi il termine «reiterate» è importante, perché qualifica in maniera più specifica la condotta che deve essere sanzionata. L'emendamento non prevede tale termine e per queste ragioni noi voteremo

Quindi, proprio accogliendo le preoccupazioni dei colleghi di non mettere a rischio l'azione del pubblico ufficiale rispetto ad interpretazioni forzose, abbiamo accolto l'emendamento del collega Di Maggio, che esplicita tale concetto. È un po' lapalissiano, perché prevedere in una norma qualcosa che già esiste nell'ordinamento vigente è ridondante, ma lo abbiamo fatto proprio per rassicurare le Forze dell'ordine. coloro che agiscono nella legittimità della norma, su mandato del magistrato, anche usando la forza, perché in quel caso è necessaria, non devono temere niente.

dunque, è stato chiesto più di una volta di spiegare: non ci dica semplicemente che è stato convinto dal buonsenso, anche perché la conoscono come persona estremamente seria e di grande libertà intellettuale. Voglio dunque capire da chi è arrivato l'ordine di cambiare quello che era stato deciso in Commissione. Lo dica con chiarezza: è stato il Governo, il commissario Lumia, o qualcun altro? Da chi ha preso l'ordine? Ce lo dica, dopodiché ci adegueremo tutti. Mi appello quindi al Capogruppo del Partito Democratico perché si faccia parte attiva e sollecita - mi pare che lo stia già facendo, visto che sta esaminando l'emendamento - per trovare una soluzione che consenta a tutti i senatori di votare in serenità un provvedimento che riguarda la tortura; si lascino perdere le supercazzole.

C'è un problema di compatibilità con la materia, ma nel momento in cui questo problema si risolve in quest'Assemblea qualsiasi senatore, indipendentemente dal fatto che in quel momento si trovi in maggioranza o in opposizione, deve essere libero di esprimersi con il proprio stile, che magari non è il mio, ma - ripeto - il suo. Questo è il principio cardine di un Parlamento libero che funziona. Non si può dare la parola a un senatore solo per associarsi, come pure è stato detto da quei banchi. Credo che questo sia qualcosa che non fa bene alla nostra istituzione.

hanno espresso perplessità sul punto specifico del provvedimento che stiamo discutendo. cari colleghi, è qualcosa che dovrebbe far riflettere tutti, perché se la perplessità viene da un settore, essa è settoriale, mentre se è generalizzata vuol dire che va al di là

avere un punto di condivisione quando abbiamo applaudito tutti quanti l'operato delle Forze dell'ordine (ripeto: lo abbiamo fatto unanimemente, senza alcuna distinzione di posizione politica o di occupazione dei posti nell'emiciclo), di fronte a una manifestazione di perplessità unanime

Sono tra i pochissimi senatori di quest'Assemblea ad avere rapporti assidui, costanti, frequenti, di confronto aperto, di discussione franca e di relazione costante con numerosi sindacati di polizia. Dunque, conosco bene perplessità e dubbi che vengono da quelle organizzazioni penso che quanto è stato prima detto corrisponda a un faticoso e spesso doloroso dibattito all'interno di quelle stesse organizzazioni. materia è infatti delicatissima, talvolta incandescente, e - dunque - produce confronto acceso e anche acute lacerazioni. Tuttavia, siamo ben lontani - lontanissimi - dall'avere un atteggiamento univoco da parte di quelle associazioni maggiormente rappresentative sul tema in questione. Dunque, una dichiarazione comune non corrisponde ad un'unità di atteggiamento; anzi. Basta avere la pazienza di ascoltare quei

sulle questioni relative a questo o quell'emendamento. Dopodiché sollevo una questione. Il Presidente, rispondendo ad un collega, ha detto ciascuno ha il suo tempo a disposizione per intervenire e che spetta poi al Presidente valutare la conformità dell'intervento alla materia e la compatibilità con quanto viene detto. Chiedo quindi al Presidente di considerare con attenzione e con il dovuto rispetto, che è proprio

gli interventi del simpaticissimo e brillantissimo senatore Giovanardi siano compatibili con la materia, nel momento in cui qualunque suo intervento prende a pretesto questo o quell'emendamento per esprimere le sue opinioni su persone che sono state vittime di gravi fatti di cronaca. Seguendo i suoi interventi abbiamo avuto, nei mesi, nei giorni e nelle ore precedenti, un elenco dettagliato di persone rispetto alle quali ci sono indagini della magistratura in corso o sentenze della magistratura già emesse o sentenze che dovranno ancora essere emesse. Per tutte queste vicende il simpaticissimo e brillantissimo senatore Giovanardi)*, sostanzialmente denigrando la figura delle vittime e, con un'esemplare manifestazione di *pietas* cristiana,

nemici dello Stato e come coloro che, alla resa dei conti, se la sono cercata. Questo vale persino per l'ultimo episodio citato stamattina, quello di Riccardo Magherini, Magherini, per il quale è accaduto quello che il senatore Giovanardi ha detto, omettendo però di ricordare che per quella vicenda, avvenuta nel marzo del 2014 a Firenze,

e garantisti pelosi, ed essendo io garantista su tutte le questioni e incondizionatamente, rispetto e approvo la sentenza della magistratura,

descritto con quelle parole brutali dal senatore Giovanardi, ieri, in un tribunale della nostra Repubblica, è stato considerato vittima di un omicidio colposo da parte di tre appartenenti all'Arma dei carabinieri. Tre e solo tre, sia chiaro. La condanna di questi tre carabinieri in primo grado, a mio avviso, non infanga in alcun modo l'onore dell'Arma, non offende in alcun modo la loro divisa, ma anzi è utilissima per dire che, se ci sono tre carabinieri responsabili di omicidio colposo nei confronti di Riccardo Magherini, ci sono centinaia di carabinieri che non sono responsabili né di illegalità, né di omicidio colposo. Un po' di equilibrio, per cortesia, senatori.

le motivazioni per cui condivide un emendamento, userà argomenti vari. Quelli usati dal senatore Giovanardi possono essere condivisi o no, ma erano tutti connessi alla materia. Dico allora al senatore Buccarella, ma con spirito costruttivo, che non è che quando voi...

sindacati delle forze di polizia e appartenenti alle forze di polizia con i quali il senatore Manconi dice di intrattenere rapporti. Anch'io, è notorio, ho contatti e rapporti, forse più graditi di quelli dell'onorevole Manconi, con queste organizzazioni. Ovviamente ha diritto di avere tutti i contatti, ma forse ha poche condivisioni.

D'Ascola. Diceva il senatore Falanga che manca la parola «reiterate», però invito il senatore Falanga a riflettere sulla seconda parte dell'emendamento, dove si dice: «Il fatto non è punibile se sono inflitte sofferenze o patimenti come conseguenza di condotte o sanzioni legittime

un esponente delle Forze dell'ordine va ad arrestare un camorrista nel quartiere di una città e i parenti si frappongono, il poliziotto, che per eseguire l'ordine d'arresto gli dà uno spintone (e fa bene, dovendo arrestare un latitante della camorra), si veda poi denunciato dal parente del camorrista come torturatore. Questa legge aiuta anche anche la camorra, oltre a mortificare le forze di polizia. mi ero augurato che nel giro di una settimana ci fosse qualche riflessione sull'argomento, ma vedo che siamo rimasti allo stesso punto della settimana scorsa.

la votazione per parti separate dell'emendamento 1.4, che, essendo composto di due periodi, viene a proposito. In particolare, il secondo periodo reintroduce ciò che aveva introdotto la Camera per quanto riguarda la tutela nel caso si tratti di sofferenze inflitte «o patimenti come conseguenza di condotte o sanzioni legittime ad esse connesse o dalle stesse cagionate».

in Commissione al Senato questo è stato soppresso nell'ambito di un accordo che, come è stato detto più volte, è stato raggiunto per dare un equilibrio al provvedimento.

che, in sede di processo, viene valutato il fatto che determinate azioni vengono condotte

giudicare se un poliziotto o un Carabiniere, in un'azione di ordine pubblico, magari fatto oggetto di lancio di oggetti, di assalti e di minacce alla propria

esimente dell'adempimento del dovere e delle funzioni pubbliche, questo poliziotto o questo carabiniere possa essere condannato. E teniamo presente

e in situazioni dove mette a repentaglio la propria incolumità. A quel punto c'è il grave rischio che subentri il ragionamento su chi glielo faccia fare. Chi glielo fa fare

ed efficace nel mio intervento. Corro un po' più lentamente, mi do da fare un po' di meno e magari un innocente rimane nelle mani del criminale, perché il poliziotto o il carabiniere, dissuaso dalle norme che qui stanno passando, tutto sommato, non ha voglia di essere di essere l'eroe che si prende la sanzione, perché poi non passa per eroe, ma per il torturatore, perché il reato si chiama tortura, non si chiama eccesso di zelo nella tutela dell'ordine pubblico. Di questo stiamo parlando e, purtroppo, come succede e non per la prima volta su questo provvedimento, si confondono e si equiparano condotte, come quelle alle quali ho accennato, con quel comportamento assolutamente odioso, riprovevole e da punire con severe sanzioni che è la tortura vera e propria.

un fatto contingente, ma scritto in questa modalità, a mio avviso, crea ancora più confusione rispetto all'intendimento del presentatore. Vorrei intervenire onestamente anche sull'ordine dei lavori, per quanto ha detto soprattutto chi l'ha preceduta

sono stati condannati a sette mesi e otto mesi, che condivido la sentenza e che non c'erano le percosse. Cinque minuti dopo il senatore Manconi mi ha accusato di non aver detto le cose che sono sul Resoconto. Quindi, sono mistificazioni continue del ragionamento svolto da chi interviene. Non sono andato io a Firenze a incidere sul processo dell'avvocato Anselmo. È stato il senatore Manconi a fare le conferenze stampa a Firenze. Io dico solo, rispettando tutte le sentenze, che quando intervengono condanne per omicidio colposo, ne prendo atto,

I tre agenti di custodia del caso Cucchi sono stati assolti, e di nuovo quest'Assemblea, come anche il Presidente della Regione Emilia, li ha citati come dei criminali. Ma, allora, quando i poliziotti sono condannati, sono colpevoli; quando sono assolti, sono colpevoli lo stesso, addirittura di tortura perché in tutto questo dibattito, caro senatore Manconi, i casi che ha citato sono anche di persone assolte non solo dalla magistratura

devo forse essere preoccupato come parlamentare di una giustizia che viene pubblicamente influenzata da persone che si vantano di costruirla tramite le menzogne,

e non mi devo indignare di queste cose? Non c'è forse odio? Scusate, se carabinieri e poliziotti assolti o condannati sono sempre colpevoli, questo cos'è? Non è un pregiudizio nei loro confronti? Io accetto le sentenze, ma per quello che c'è scritto:

signor Presidente, resto molto stupito per la richiesta del senatore Orellana che vuole addirittura il contingentamento dei tempi, quando appare del tutto evidente che c'è una tattica dilatoria dei tempi in corso, perché alcuni Capigruppo di maggioranza e qualcuno di opposizione si sono appartati con il relatore per trovare evidentemente una quadra su un emendamento che altrimenti avrebbe difficoltà a essere digerito. È una dinamica parlamentare legittima, corretta, ma sarebbe meglio se fosse fatta in Commissione, o quantomeno se ci fosse una circostanza che consentisse a tutte le parti di partecipare a questa dinamica. Credo, Presidente, che non sfugga alla sua attenzione la necessità di ritrovare serenità nella gestione di questo provvedimento, perché anche i termini che scaturiscono dal dibattito sugli emendamenti dicono che si sta rischiando, ogni volta, di cascare

Presidente, anche l'emendamento 1.202 meriterebbe, a mio avviso, una votazione per parti separate.

quando le sofferenze fisiche o psichiche derivano unicamente da sanzioni legittime, sono ad esse inerenti o da esse provocate». Ebbene, questa seconda parte mi pare possa essere condivisa da tutta l'Assemblea. Se la sofferenza non è causata da una condotta di percosse o quant'altro, da parte di chicchessia, ma è la causa diretta della sanzione

affidando il proprio linguaggio anche ad aggettivi che attengono alle caratteristiche della persona alla quale risponde, e poi che cosa fa? Va via e non aspetta che altri gli diano risposte in ordine alle sue affermazioni. Rispetto molto il senatore Manconi, ma egli abbia rispetto e non si

Presidente, mi dispiace parlare parzialmente in disaccordo con il senatore Manconi, dal momento che ho sempre condiviso con lui due linee: prima è quella di credere che non siano necessarie pene più alte per creare deterrenza, la seconda è che non credo nell'uso della forza, per il principio fissato all'articolo 2 della Costituzione. Per la dignità della persona umana, l'uso della forza, anche quando è legittimo, va limitato,

la Camera aveva introdotto una giustificazione ben più forte dell'uso legittimo della forza.

si era posta il problema di come evitare la possibilità che le azioni delle forze di polizia fossero condizionate dalla paura di incappare in un procedimento penale: non un procedimento penale dal quale venir condannati, ma dal fatto che sia iscritto.

che pure condivido, nel momento in cui afferma che vi è una violazione delle funzioni o l'abuso del diritto. Per quanto riguarda il testo approvato dalla Camera vi era una limitazione ulteriore. In Commissione,

e dava la possibilità che la forza di polizia non fosse preoccupata. Ciò non toglie che, invece, se ci fossero state delle azioni sbagliate, queste avrebbero dovuto essere colpite, giudicate, individuati i responsabili e condannati.

quindi, un'attenzione molto forte: non è una questione di difesa corporativa di interessi, non vi è una posizione politica tale da non dover essere condivisa. Ripeto: la mia posizione parte da quella del senatore Manconi, come concetto e come decisione, però dove arriviamo? Qual è il risultato? Io voglio che la forza di polizia che commette una semplice lesione sia punita e condannata per lesioni; se invece commette le ipotesi che sono configurate in questo testo deve essere condannata per tortura.

Ve lo dico sinceramente: non sono riuscito a capire la ragione per la quale eliminare la parola «reiterate» proposta da uno dei relatori, il presidente D'Ascola, e votata da tutti noi. Qual è la ragione? Ho molto apprezzato che non tutto il Partito Democratico abbia presentato emendamenti. Ho molto apprezzato che gli altri si siano attenuti a quella regola.

per cui, se il poliziotto ha commesso abuso dei poteri oppure ha determinato alcune situazioni non corrette da un punto di vista delle proprie funzioni, in quel caso non è punibile.

dobbiamo stare attenti a non creare allarmismo nelle forze di polizia, dobbiamo stare attenti a non creare una situazione di preoccupazione di essere iscritti nel registro degli indagati. È questa la ragione che vi rassegno e addirittura invito il collega Di Maggio a ritirare il proprio emendamento, se viene mantenuto il «reiterate», perché questo significherebbe dare un equilibrio maggiore all'intero sistema dal punto di vista tecnico-giuridico. Avete dei consulenti, presidente Zanda, dei professori di diritto penale: chiedete loro se è corretto quello che sto dicendo oppure no.

e si informi dai suoi esperti e consulenti se è corretto quello che ho detto. Avete professionisti di diritto penale come il collega Cucca e altri: domandate qual è la ragione.

Dobbiamo condannare chi commette questi fatti? Certamente sì. Dobbiamo evitare che le forze di polizia siano bloccate dalla preoccupazione? Certamente sì. Tra queste due affermazioni passa un equilibrio che era stato raggiunto in Commissione.

allora una risposta: io dico che è un comportamento legittimo quello delle forze dell'ordine che fermano e bloccano una persona, un violento, un assassino, uno stupratore,

«reiterate» serviva a dire che i carabinieri che hanno bloccato il potenziale assassino non ricadono

e quindi c'è una colluttazione, nel momento in cui entrerà in vigore questa norma, ci sarà per tutti loro una denuncia e quindi un processo di anni, uno spostamento di sede, un trauma per i figli, una canea mediatica, il solito circo mediatico che girerà per tutta l'Italia a dire che loro sono assassini.

Commissione abbiamo detto che se l'Europa ce lo chiede, perché non introduciamo immediatamente la norma europea sulla tortura? È chiarissimo quello che dice la norma europea: la tortura è il caso Regeni. Quello sì, si capisce benissimo che è un caso di tortura. Quello che stiamo introducendo non è tortura,

Signor Presidente, nel corso di questa discussione, fermi restando ovviamente i legittimi convincimenti degli onorevoli senatori, vorrei solo ribadire a nome del Governo che non vi è, da parte nostra, nel parere favorevole all'accoglimento dell'emendamento in esame, alcuna indicazione che possa in qualche modo ledere non solo la sicurezza, ma anche l'autonomia delle Forze dell'ordine. Si tratta di una norma che chiarisce, sulla base di una interpretazione che è stata qui già fornita dal presidente della Commissione D'Ascola, quale sia il contesto entro il quale si verifica la condizione della tortura, Non farò qui il catalogo degli esempi concreti, che ovviamente appartengono alla discussione dei singoli senatori, mi pare altrettanto importante segnalare che questo reato è previsto in condizioni particolari di privazione della libertà non può avvenire all'interno di circostanze che vedano un conflitto tra le Forze dell'ordine e i soggetti che potrebbero eventualmente reagire. Si tratta di una una precisazione che, peraltro - e anche questo è molto importante dal nostro punto di vista - raggiunge un equilibrio sulla base delle diverse formulazioni che sono state successivamente indicate dalle Assemblee e dalle Commissioni,

non è che dobbiamo timbrare il cartellino e produrre una quantità di leggi. Questo è un punto delicato: stiamo discutendo - lo dico con molta pacatezza - della possibilità di intervento delle forza di polizia e delle Forze dell'ordine, di quando è legittimo

forze di polizia.

di tesi favorevoli alla mafia o a cosa nostra; egli sostiene un punto di vista critico perché, nella sua posizione garantista a 360 gradi, ritiene - più volte ho letto suoi interventi in tal senso

Ha detto Renzi che rinnoverà loro il contratto, che però non è stato ancora rinnovato. Speriamo che lo rinnovi, oltre agli 80 euro, per consentire loro di pagarsi le spese legali, che probabilmente cresceranno, perché aumenteranno le possibilità di denuncia per presunte torture. Ho fatto prima l'esempio dell'arresto di camorristi e di mafiosi: quante volte quartieri o Comuni interi sono

proprio al fine di bilanciare il contenuto di una norma. Ricordo che è stata proprio la Commissione a togliere l'inciso che era stato varato dalla Camera e che diceva che, ai fini dell'applicazione del primo e del secondo comma, la sofferenza deve essere ulteriore rispetto a quella che deriva dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.

e pensiamo: questo disegno di legge e nello specifico questa norma, per come la volete introdurre, dove prevede quelle condotte degradanti per la dignità umana? Dove vengono inserite quelle ipotesi che riguardano quelle particolari forme di maltrattamento e quelle ipotesi di trattamento degradante? Dove Dove è qui il reato di tortura? Non c'è alcuna differenza tra una condotta di violenza o di minaccia grave, perché non prevede nient'altro che un tipo di evento, ovvero l'aver provocato una sofferenza fisica o un trauma psichico.

comunque non cambia il contenuto di una previsione che noi non condividiamo, ma almeno la parola «reiterate» serviva a bilanciare un sistema.

vede una parte del Parlamento poco favorevole, dunque non voglio contribuire anch'io con i miei interventi a rendere la discussione ancora più complessa. Ho l'impressione che vi sia un punto

per attuare nell'ordinamento giuridico del nostro Paese una convenzione internazionale, che peraltro risale al 1984. E pensiamo - per questa ragione, ripeto, abbiamo presentato questo emendamento che evidentemente il criterio guida, nel momento in cui si applica e si attua nel nostro ordinamento giuridico una norma prevista da una convenzione internazionale, debba essere quello della massima conformità del nostro testo al testo della convenzione stessa. Noi crediamo che le modifiche apportate al testo

Riterremmo, evidentemente, molto sbagliato se il Parlamento, approvando una norma differente da quella prevista dalla Convenzione, desse una interpretazione tutta italiana. italiana. Dico ai miei colleghi che tutti i Paesi del mondo che hanno applicato la Convenzione hanno parlato di tortura esattamente nei termini che sono stati discussi dall'ONU addirittura nel 1984. L'anomalia

Presidente, senatrici e senatori, intervengo per sgombrare il campo da una possibile fonte di equivoci, anche pesante, e per fare chiarezza. Ho apprezzato come il senatore Gasparri abbia esposto le sue critiche alle posizioni da me espresse sul regime del 41-*bis*. È importante precisare che, al di là delle mie posizioni personali,

massimamente apprezzato, con parole addirittura lusinghiere, da giuristi come Gherardo Colombo e Giovanni Maria Flick, mai, neanche una volta, quel sistema e quel regime vengono assimilati alla tortura. Non c'è mai una sola formula, una sola parola che possa produrre un tale equivoco.

fine, interrompere e non consentire in alcun modo la prosecuzione delle relazioni tra le persone detenute sottoposte al 41-*bis* e la criminalità esterna. Questo è lo scopo, il fine esclusivo Noi, dunque, abbiamo valutato l'applicazione di quel sistema solo ed esclusivamente attraverso questo criterio e questo indicatore, rilevando come spesso, nell'applicazione concreta a quello scopo esclusivo del regime di 41-*bis*, si aggiungano poi afflizioni, inutili restrizioni, limiti imposti che, ovviamente, risultano illegali perché non contemplati dalla norma che prevede il 41-*bis*. Dico però con serenità, perché non c'è dubbio su questo, che mai, in alcun momento di quel rapporto, si assimila il regime di 41-*bis* al delitto di tortura. Questo è per fare chiarezza e perché la nostra discussione non sia condizionata da fattori che possano inquinarne la chiarezza assoluta e l'atteggiamento di ciascuno di noi.

Grazie di comportarsi con il tipico atteggiamento del tifo calcistico: tanto più autorevoli saranno le nostre decisioni, quanto meno ci si schiererà su diverse contrapposizioni e fazioni.

tutta la fase istruttoria all'interno della Commissione - vi sia il tentativo necessario di trovare dei punti di equilibrio.

devo dare atto che i relatori e il Presidente della Commissione hanno contribuito al tentativo di trovare un punto di equilibrio, che evidentemente in Aula porta momenti di esasperazione. quel momento essenziale che una norma come quella in esame richiede e del quale ha bisogno. Dobbiamo colmare una lacuna che - come giustamente sosteneva il senatore De Cristofaro - è ormai datata al 1984 ed è l'individuazione del reato di tortura all'interno del nostro ordinamento.

Quindi, la fatica di trovare un equilibrio, affinché non ci siano posizioni da tifo calcistico, mi sembra doverosa. Ricordo poi al collega, senatore Gasparri, che l'emendamento che la Commissione ha approvato e che mi ha chiesto di ritirare non è poi così tanto una foglia di fico, se lo stesso emendamento 1.202, che lei ha presentato, prevede esattamente la stessa cosa che ho chiesto io con il mio. Quindi, non credo sia una foglia di fico, ma ritengo vada a tutela delle Forze dell'ordine, che - come molto spesso è stato spiegato in quest'Aula - vedono in questo provvedimento qualcosa che possa censurare il loro comportamento. Credo che non sia così e che l'animo del legislatore sia di prestare ulteriori garanzie: questa è anche l'ottica e il senso dell'emendamento che ho presentato.

probabilmente non in perfetta sincerità e onestà intellettuale, si vuole ergere in quest'Aula come difensore delle Forze dell'ordine: atteggiamento rispettabilissimo, ma forse meno rispettabile, almeno da parte di chi parla, quando non sussiste un ragionamento

auspicabilmente per l'ultima volta nel passaggio in questo ramo del Parlamento - è un reato cosiddetto comune; non è un reato proprio, non è un reato dei poliziotti e dei carabinieri, ma fortunatamente - come abbiamo sempre sostenuto - potrà interessare chiunque porrà in essere quei comportamenti che abbiamo cercato di definire come tortura, nella piena consapevolezza della complessità che ciò comporta, perché qualsiasi testo si possa provare a elaborare potrà sempre essere oggetto di critiche più o meno fondate. Vorrei fare un invito ai colleghi senatori che esprimono queste perplessità: proviamo a pensare alla prossima volta - senza voler andare indietro nel tempo - in cui accadranno quegli episodi drammatici e odiosi, come per esempio le rapine in villa, l'anziano imprenditore veneto, lombardo o siciliano, sarà sequestrato in casa, legato, sottoposto a tortura, magari per avere la combinazione della cassaforte. della cassaforte. Avrete il coraggio di sostenere che una semplice tortura - perché non reiterata - fa sì che quel reato non sussista? Non pensiamo solo ai poliziotti o ai carabinieri: pensiamo a mafiosi, ai rapinatori, e a tutte le volte in cui le argomentazioni di chi vuole mantenere

extra comunitario - mettiamoci anche l'aggravante - che sequestra e sottopone a tortura un cittadino italiano, o straniero a sua volta, pur non essendo poliziotto. Sarà necessario prevedere la reiterazione delle torture? Non basterà il taglio di un orecchio? Non basterà un *waterboarding* fatto a casa nel tinello per dire che è tortura? Colleghi, abbiate allora un po' di onestà intellettuale e andiamo avanti velocemente.

tutti gli istituti che fanno indagini demoscopiche, Sottosegretario, ci dicono che i cittadini, quando viene richiesto loro in chi hanno fiducia, rispondono Carabinieri,

Questo è il motivo del mio intervento. Voglio stare con i cittadini, senza se e senza ma, come il Gruppo di Forza Italia, dalle parte delle Forze dell'ordine. I cittadini ci dicono che fanno un lavoro di cui dobbiamo ringraziarli ogni giorno; ci sono martiri ed eroi, e questa non è retorica. Ma se il Capo della Polizia ci dice che quello che facciamo non va bene; se le Forze dell'ordine lanciano

che gli interventi che vengono svolti dalle Forze dell'ordine sono per il 90 per cento delle volte di emergenza. E voi pensate che le persone che vanno ad arrestare, su cui devono intervenire in flagrante, e da cui spesso devono difendersi, non useranno poi questo

che io, il senatore Fazzone, chi ha avuto modo di frequentare fortemente le Forze dell'ordine, siccome in esse crediamo, ci rifiutiamo di pensare che il Senato della Repubblica possa votare contro di loro, e per questo non parteciperemo al voto.

Presidente, la piega che sta prendendo la discussione mi porta ancora una volta a chiedere di sospendere la seduta e di verificare con maggiore serenità il contenuto degli emendamenti, e soprattutto come poi gli stessi vengono interpretati. Quanto detto dal senatore Buccarella poco fa è nettamente in contrasto con l'opinione espressa prima dalla senatrice Stefani, piuttosto che da me, pur essendo lo stesso tipo di emendamento. È evidente che, nel momento in cui si inserisce nel provvedimento un avverbio, un aggettivo o una formula, lo stesso, a seconda di come lo si guarda, può essere interpretato a favore o contro le Forze dell'ordine,

Io vorrei veramente che non ci fosse da parte di qualche senatore l'intenzione di equiparare l'azione legittima che svolge con difficoltà un tutore delle Forze dell'ordine rispetto invece a quella di un criminale che si comporta come tale nei confronti di gente che subisce il crimine. Non è la stessa cosa. Non possiamo equiparare questi due elementi. Non possiamo equiparare il carabiniere, l'agente di polizia, un rappresentante delle Forze dell'ordine

nei tutori delle Forze dell'ordine e nei cittadini circa da che parte sta lo Stato. È ora di finirla con queste cose. E mi rivolgo anche al Governo. Fermatevi, fermiamoci, mettete i puntini sulle i e date un senso a questo provvedimento che non deve essere un qualcosa di ambiguo o di equivoco che rischia addirittura di equiparare l'agente di polizia, un rappresentante delle Forze dell'ordine a un criminale che sta commettendo un crimine.

si è fatta una certa fatica e ne è uscito un mezzo pasticcio nel cercare di stabilire quale sia il confine tra il reato di tortura propriamente detto e l'abuso delle prerogative dell'uso legittimo della violenza,

a distinguere i momenti in cui effettivamente degli abusi sono stati svolti in passato da parte delle forze di polizia e i momenti in cui invece sono state fatte delle speculazioni e strumentalizzazioni sui comportamenti delle stesse forze di polizia. Tanto per essere chiari, io sono di quelli che ha presentato un'interrogazione sul caso Magherini, di cui si è parlato oggi. Non si può, però, sentire dire qualunque cosa. È evidente che la norma che stiamo discutendo

presenti tutte le aggravanti possibili (l'omicidio volontario). E non è certo il reato di tortura che cambierà la qualità della vita del proprietario della villa, dei suoi eredi o parenti.

ed è evidente che, nel caso di specie, la norma in questione non mi convincerebbe minimamente neppure se ricomprendesse il termine «reiterato». che in ogni caso quel reiterato tendeva a stabilire una delle caratteristiche specifiche del reato di tortura. È certo, infatti, che la tortura non è una violenza occasionale esercitata nei confronti di una persona che non è in condizioni di libertà.

È questa la ragione per cui le forze di polizia la valutano con grande preoccupazione. Ed è la ragione per cui io, nonostante presti una grande attenzione rispetto alla necessità di sanzionare gli abusi posti in essere (soprattutto in alcuni anni storici particolarmente difficili di questo Paese) da parte delle forze di polizia, non posso però negare l'evidenza di essere di fronte a un testo che sostanzialmente - peraltro in un contesto storico completamente mutato - chiude la stalla dove sono scappati i buoi; e soprattutto la chiude male, perché crea oggettivamente una serie di problemi enormi sui rischi professionali nello svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria nel nostro Paese.

una proposta e, se si vuole, un appello all'Assemblea. Viste le condizioni del nostro lavoro e dato che in realtà manca vorrei riprendere con forza e con spirito costruttivo l'invito venuto dal senatore Candiani a operare una sospensione che sia in qualche modo anche una ricerca vera ed effettiva di una soluzione, tenuto conto che il dibattito di oggi è stato sicuramente lungo ma ricco e si è svolto nel merito. Io credo tutte le forze politiche hanno il dovere di tentare di arrivare su questo punto alla maggioranza più ampia possibile. Ovviamente non c'è alcuna certezza che ciò possa avvenire, ma io credo anche che inviti ad andare avanti e a fare presto, se sono legittimati da una ricerca effettiva di soluzioni di consenso, vista la materia, potranno magari avere più forza alla ripresa dei nostri lavori. Chiederei quindi alle forze di maggioranza ed alla maggioranza occasionale che si verrebbe a formare

Presidente, io credo che il Parlamento - e il Senato, naturalmente - abbia un debito con la società italiana e con l'ordinamento internazionale e che questo debito debba

le richieste di rinviare la decisione non possano essere accolte. Credo che noi tutti dobbiamo tener presente quali sono le condizioni nelle quali siamo arrivati finalmente a

Siamo arrivati alla seduta di questa mattina dopo aver già ampiamente usato molto del nostro tempo, anche nelle sedute precedenti. Ora stiamo discutendo di una questione specifica e, se permettete, con tutto il rispetto nei confronti delle varie opinioni che sono state espresse, il dibattito di Aula non ha favorito finora la chiarezza e l'intelligenza del problema di cui stiamo parlando. Infatti, conversando con molti colleghi,

non era chiara perché - lo ripeto, come ho già detto altre volte - il dibattito d'Aula è difficile, è molto complicato. Il dibattito d'Aula che mischia posizioni politiche a posizioni di merito rende ancora più difficili questioni che già lo sono di per se stesse. È chiaro che, se arriviamo con vent'anni di ritardo a introdurre un reato rispetto al

È in gioco, naturalmente, il diritto dello Stato a far valere, anche con la forza, la legge. È un diritto fondamentale, senza il quale le democrazie non possono sopravvivere.

l'utilizzo di strumenti che possano essere definiti di tortura - e mi sembra che la formula che è stata proposta, di cui ora stiamo discutendo,

cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà (...)». E lo sottolineo. Parliamo di «violenze», «minacce gravi», «agendo con crudeltà», «cagiona (...) sofferenze fisiche» a una persona che è privata della libertà personale. Voi capite che in una democrazia questo è comunque inaccettabile. Questa formula ha avuto una ha avuto una vita, una storia. La Commissione la sta esaminando da più di due anni, senza ricordare quando l'ha esaminata nelle precedenti legislature. Il termine «reiterate» è comparso e scomparso. La Commissione ha approvato in una prima fase una versione nella quale l'espressione «reiterate violenze» non compariva.

nelle leggi le parole debbono essere misurate ed è dannoso aggiungerne inutili - era assolutamente inutile aggiungere la parola «reiterate».

Abbiamo dei provvedimenti molto importanti da esaminare. Francamente penso che l'importanza del tema, l'approfondimento fatto e la consapevolezza che ormai tutti i senatori hanno del problema rendano necessario votare.

calibrare in maniera corretta ed equilibrata la doverosa tutela dei cittadini, a cui lei faceva riferimento,

parole «minacce» e «violenze» configura la fattispecie delittuosa solo quando vi sono più condotte minacciose e violente,

molto spesso delle difficoltà di interpretazione alla magistratura e agli organi giudicanti: uno in più Presidente Zanda, ancorché lei dica che non vi è un significato politico in una maggioranza, che questa mattina, su tale questione, si realizza tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle,

fu eliminata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, perché al Senato, in prima lettura, abbiamo redatto e stilato la norma

diritto. Caro presidente Zanda, per rafforzare quell'equilibrio tra le due posizioni che dobbiamo calibrare, chiediamo che ci siano una maggiore incidenza e una maggiore qualificazione del delitto di tortura, perché si realizza con ciò quella calibratura che - a nostro avviso - è necessaria tra la tutela dei diritti del cittadino, a cui tanto il presidente Manconi fa spesso riferimento, e la tutela dell'operatività delle Forze dell'ordine. Se ciò è inutile, così come dice il presidente Zanda, mi domando perché mai oggi si rifiuta, per qualcosa di inutile, l'appoggio del mio Gruppo in questa Assemblea, che non è mancato in altri momenti e che non mancherebbe neanche oggi. Ma noi non siamo disponibili a realizzare quell'intendimento tenebroso, oscuro, antipatico e odioso di accettare quando servono e di non accettare e non gradire quando non servono. Questo ci sta stancando, siamo stanchi di questo modo di fare. È per questa ragione che, condividendo le argomentazioni del senatore Quagliariello, di dire, signori cari, che non è vero che non c'è una valenza anche politica. Riflettete, perché domani le nostre dichiarazioni e i commenti della stampa potranno lasciar immaginare alla pubblica opinione ciò che forse è vero: una maggioranza diversa in questo Senato della Repubblica. *(Applausi del senatore Quagliariello)*. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire solo per confermare che accolgo la proposta

opinioni. Non ci stiamo perché tutte le volte che il dibattito parlamentare va oltre i tempi che voi avete previsto, dei capigruppo, dove voi fate le vostre proposte, intervenite e ci impedite di trattare, parlare e far capire anche a chi sta fuori quali sono le posizioni dei vari Gruppi parlamentari e dei singoli parlamentari.

è scandaloso nei confronti di tutti gli uomini e le donne delle forze di polizia che, oggi come oggi, fanno i salti mortali per mantenere l'ordine pubblico in questo Paese. Quindi noi non vogliamo punire le Forze dell'ordine, noi non vogliamo limitare le Forze dell'ordine, noi non vogliamo sentir dire che d'ora in poi le Forze dell'ordine non possono più fare quello che vogliono. Non lo vogliamo sentire, perché le Forze dell'ordine stanno mantenendo l'ordine pubblico in questo Paese,

chiede una società diversa rispetto a quella che state portando avanti voi, rispetto allo schifo di questo Paese. Basta leggere i giornali o ascoltare la televisione per vedere quello che succede.

Chiedete la fiducia, così almeno la finiamo lì *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*, e così almeno fuori, ancora una volta, vedranno da chi è composta questa maggioranza. Questa è una maggioranza ormai variabile sugli argomenti, in cui chi è seduto alla mia destra fuori parla bene e dentro razzola male. E finalmente anche i cittadini vedranno cosa fanno i colleghi alla nostra destra.

informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione».

Vorrei far presente che la Convenzione di New York dice cose totalmente diverse da quelle di questo disegno di legge. Se la Convenzione di New York fosse recepita immediatamente dal Parlamento italiano, a me andrebbe benissimo, perché cos'è la tortura e cosa viene definito tortura: estorcere confessioni, estorcere informazioni, discriminazioni di cui è fatta oggetto la persona. Ciò è assolutamente lontanissimo dal testo di cui stiamo discutendo. Coprirsi con una convenzione internazionale per introdurre concetti totalmente diversi non è onestà intellettuale, perché - ripeto - basterebbe introdurre nel nostro ordinamento la Convenzione di New York ed avremmo già risolto il problema dei nostri ritardi. Ma dico di più al senatore Manconi.

Caro senatore Manconi, intanto mi aspetto che lei mi dia atto della mia onestà intellettuale, visto che lei ha detto che il senatore Giovanardi non ha ricordato che sono stati condannati. Sono stati condannati a sette mesi per omicidio colposo, perché non hanno previsto che tenere quel signore in quella posizione poteva provocare, visto che era strafatto di cocaina, una certa conseguenza. Detto ciò, veniamo al sodo. Per me quei carabinieri hanno delle esimenti, mentre il giudice li ha condannati per omicidio colposo, ed io lo accetto; ma per metà di quest'Aula è tortura, perché è una settimana che sento dire da Presidenti di Regione e da colleghi in quest'Aula che quell'episodio dei tre carabinieri è tortura, quindi dovrebbero andare all'ergastolo.

dove può capitare - ahimè - che qualche volta siano assolti perché non hanno fatto niente, ed altre volte che sia omicidio colposo perché c'è stata negligenza. Tutta la discussione delle forze politiche in quest'Aula è per designare come tortura da punire con l'ergastolo questo intervento dei poliziotti e dei carabinieri, dove non c'è alcuna traccia della tortura di cui parla la Convenzione internazionale. Presidente Zanda, di questo stiamo parlando. Mi spieghi allora dove la Convenzione internazionale si applica alle norme scritte in Commissione. Mi dica perché non recepiamo nel nostro ordinamento il testo della Convenzione di New York sulla tortura: a me starebbe benissimo, perché si colpisce la vera tortura, come ha detto il collega Augello, e non cose diverse che non hanno niente a che fare con la tortura. È evidente che c'è un pregiudizio verso le Forze dell'ordine grande come una casa, perché si vogliono criminalizzare comportamenti colposi, non dolosi. Qui si parla di atteggiamenti, in tutti i casi che abbiamo citato (che sono i casi di scuola che vengono ripetutamente citati anche dal senatore Manconi), al limite della negligenza e dell'imperizia, non di reati dolosi condannabili fino all'ergastolo.

indicato come colpose (e continuava ad insistere sulla colpa e sulla criminalizzazione anche quando gli agenti erano stati assolti). Continuano ad essere riportati i nomi di questi agenti pienamente assolti, che non avevano alcuna responsabilità, come torturatori e come assassini: andate a vedere sui *social network*. E queste cose trovano cassa di risonanza in Parlamento. Noi stiamo parlando della tortura e vogliamo introdurre il reato di tortura, mentre voi state lavorando su una fattispecie ideologica che criminalizza

Colleghi, qui l'unica cosa certa è che il Regolamento lo conosco e lo applico. Il senatore Giovanardi è intervenuto in dichiarazione di voto, è poi intervenuto il sottosegretario Migliore, ed un senatore per Gruppo per dieci minuti può intervenire.

Il testo che stiamo trattando, cioè il primo articolo che definisce il reato, non prevede un reato specifico per le Forze

un atto che corrisponde a questa fattispecie, vedranno applicata un'aggravante, come previsto nel nostro ordinamento ogni volta che le Forze dell'ordine commettano un reato che è punito per tutti i cittadini. Quindi, l'articolo di cui lei sta parlando

La fattispecie del primo comma si applica al pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Quindi, per valutare quale sia il comportamento rilevante del pubblico ufficiale ai fini dell'aggravante si deve tenere conto di quanto descritto al primo comma.

perché la questione da lui posta era talmente evidente che, nel corso del dibattito, ne avevamo discusso tutti. Ricordo, tra gli altri, gli interventi del senatore Buccarella e del sottoscritto. È a tutti noto che questa legge

Quindi questo provvedimento non c'entra niente con quello che la Convenzione ci impone di fare. Non c'entra niente con la tortura come è stata indicata a livello internazionale. Stiamo introducendo nel nostro ordinamento una spada di Damocle davanti a tutti i carabinieri e poliziotti che non che voglia dare loro un suggerimento - avranno dei bei problemi quando, in difesa di 60 milioni di cittadini italiani che si trovano in difficoltà e li chiamano per aiutarli, sapranno che, per volontà di questo Parlamento e di questa maggioranza, il loro intervento, se succede qualcosa di fortuito e non voluto, può portarli all'ergastolo o comunque a un processo che dura anni, con il solito circuito di persone che girano l'Italia per criminalizzarli e per fare conferenze stampa, con tutti gli avvocati Anselmo e quello che abbiamo visto in azione in questi anni, per portare a una criminalizzazione preventiva delle Forze dell'ordine ogni volta che intervengono. a dire - bastava introdurre la norma internazionale nel nostro ordinamento e avevamo già risolto il problema. Tutti sapevamo che la tortura era quella. Tutti sappiamo - anche nell'immaginario collettivo - cos'è una tortura: quando una persona, cui è tolta la libertà, viene messa lì e viene sottoposta a pressioni fisiche e psicologiche di ogni tipo, con l'acqua, inducendo

o allo schiaffo, perché durante una colluttazione basta che uno per due volte un agente dica a un delinquente «fermati», «fermati o ti arresto», «fermati o ti sbatto in galera», «fermati o ti rovino»

nel registro degli indagati, dopodiché andranno sotto processo e verrà chiamato un perito il quale dovrà stabilire se effettivamente il trauma psichico ci sia stato o no. E questa sarebbe la tortura della Convenzione di New York? E questo sarebbe quello che succede nei Paesi del Terzo mondo, dove prendono le persone, le sequestrano, le tengono per giorni e sono sottoposte alle efferatezze e alle sevizie più terribili? Questo è paragonabile alle fattispecie di cui abbiamo parlato? Adesso non rifaccio tutta la cantilena dei nomi, ma siete stati voi a farla. Siete voi, a tutti i livelli, compresi i vostri Presidenti di Regione, a tirare fuori come una cantilena questi nomi a criminalizzare la Polizia per fatti semplicemente colposi che voi trasformerete nel reato di tortura. Questo emendamento almeno con «gravissime e reiterate», perché - come è stato giustamente ricordato dai colleghi che sono intervenuti - dalla Diaz fino agli altri casi le condanne ci sono state: state: abbiamo le percosse, abbiamo l'omicidio colposo, abbiamo tutta una serie di comportamenti che vengono, giustamente o ingiustamente - a seconda dei punti di vista, a seconda anche della persona e dell'opinione pubblica - sottoposti a sanzioni penali. oltre a questo, qui si aggiunge invece una fattispecie che porta all'ergastolo. Per la centesima volta faccio la domanda, ma la farò anche fuori, all'opinione pubblica, raccogliendo consensi: i carabinieri che davanti a Palazzo Chigi hanno fermato quello che ha cercato di ammazzare un collega sono degli eroi

sindacati di Polizia che raggruppano il 90 per cento degli agenti, scrivere cose terribili su questo provvedimento. Non so lui, presidente di una Commissione, con quale sindacato di polizia stia parlando, perché quelli con cui ho parlato io sono tutti maggioritari, di centrodestra e di centrosinistra: rappresentano tutto il

Come ho detto all'inizio, prima si tutelano i cittadini che vengono aggrediti dalla criminalità, poi le Forze dell'ordine che devono intervenire mettendo a rischio la loro vita, poi giustamente anche i criminali: le persone che commettono reati devono essere tutelate, ma in quest'ordine. Non possiamo invece cambiare l'ordine per cui prima vanno tutelati i criminali, poi eventualmente i cittadini e poi magari le Forze dell'ordine. A me sembra veramente una cosa surreale. Vorrei vedere un dibattito di questo tipo al Congresso degli Stati

perché usano le armi solo quando sono tirati per il collo, molte volte troppo tardi. Per chi va alle feste della Polizia e dei Carabinieri è molto triste sentire il rullo di tamburi e vedere le vedove,

naturalmente avendo tanti clienti, perché è bravo - che lui è in grado, condizionando i *media*, la televisione, la radio, e il TG3, di vincere i processi. Vi rendete conto a che punto siamo arrivati?

le sentenze. Non è che non le accetto: posso condividerle o no, ma le accetto. È l'altra parte che, quando le sentenze finiscono con l'assoluzione, non le accetta e continua a dire che carabinieri e poliziotti sono comunque degli assassini.

ha mostrato insofferenza per alcuni interventi; colleghi, fate male, perché c'è un tempo per la discussione e c'è un tempo di votazione, quindi credo sia giusto soppesare le parole e valutare tutto. Io sono molto amareggiato per il voto di poco fa,

anche prevedendo una seconda parte che chiariva in maniera molto esplicita la limitazione dell'applicazione di queste norme a chi faceva un uso legittimo della forza. Gli emendamenti vanno quindi intesi nella loro interezza; si poteva anche togliere la parola «reiterate» e inserire altri criteri tesi a evitare una presunzione di colpa nei confronti di chi fa un uso legittimo della forza. Tuttavia, il dibattito di questa mattina e la votazione di poco fa hanno introdotto un elemento di chiarezza, cari colleghi.

con puntualità dai senatori Caliendo e Giovanardi, gli emendamenti della senatrice Stefani sono chiari, come lo sono anche le posizioni espresse nei giorni scorsi dal senatore Palma, con la competenza di persona che ha vissuto parte della sua vita immerso nelle fonti del diritto e nella loro applicazione. Insomma, abbiamo spiegato chiaramente che il testo si doveva votare con modalità diverse. Abbiamo anche visto un dibattito tra di voi. Infatti, senatore Esposito, qualche no TAV - quelli che usano le balestre e le biglie contro le forze di polizia - magari dirà

non è una cosa che si possa fronteggiare con un'ondata di *e-mail*. Diranno: «Ci hanno torturato!» e io so che molti colleghi dello schieramento a me avverso politicamente - ma certo non nemico, siamo avversari

e le biglie in piazza Alimonda, dove il questore gli dice che non deve andare (colgo così l'occasione per solidarizzare con uno dei vari sindacati). Penso che sostenere questo emendamento e gli altri (tra l'altro, comunque oggi il provvedimento non sarebbe concluso, quindi possiamo anche soppesare meglio le ragioni di quell'emendamento nella seduta successiva) sarebbe stato un atto di saggezza. È vero, come ho detto prima, che si può cambiare in Assemblea ciò che si è deciso in Commissione (ci mancherebbe, altrimenti cosa ci stiamo a fare), tuttavia quando il cambiamento è importante e delicato forse un momento di riflessione sarebbe utile. Sappiamo che la Commissione giustizia è sempre portatrice di dubbi, perché

Signor Presidente, mi permetto di ricordare a quest'Assemblea il concetto di gravità. Cos'è la gravità? La gravità è una componente oggettiva della condotta e, in quanto tale, è ponderabile dall'esterno.

significa sostanzialmente affidare alla dimensione soggettiva tutte le prevedibili conseguenze in tema di certezza del diritto. Il requisito della gravità - lo ricordo in particolare al Sottosegretario presente in Aula - è un concetto già ampiamente presente e noto nel nostro sistema penale. Si pensi, ad esempio, alle minacce gravi di cui all'articolo 612, secondo comma, del codice penale. Appare, quindi, importante connotare questa fattispecie delittuosa

di eliminare la parola «grave» già mi pare essere stata un'operazione - lo ripeto - non curata e governata da un operatore del diritto, ma piuttosto da altri esercenti, con tutto il rispetto per le diverse professioni. Oggi, il senatore Lo Giudice mi pare abbia

furbizia di riformare il proprio emendamento denota una disonestà intellettuale e politica,

Signori, questi giochetti vanno bene, li comprendo e, forse, sono anche disponibile a praticarli, ma non su un tema così delicato come il reato

di un provvedimento su questo tema. Le obbligazioni si adempiono, si pagano, ma non con monete false. Presidente Zanda,

l'elemento oggettivo, esterno alla norma e ponderabile, che vincola

nel senso che votiamo ciò che condividiamo e non votiamo ciò che non condividiamo. Senatrice Stefani, la ringrazio per questo emendamento e mi dispiace, creda, che apprezzato da me, non sia stato apprezzato dagli altri.

Signor Presidente, il 23 settembre 2015, insieme al senatore Manconi, a seguito del tentativo di suicidio di un detenuto del carcere di Modena, che mesi prima aveva fatto istanza di detenzione domiciliare

l'ufficio di sorveglianza di Modena e, in questo caso, quali interventi intendesse adottare per porvi rimedio. Nessuna risposta. Intanto, la situazione si è aggravata. Il 13 e 14 luglio il Coordinamento regionale delle Camere penali dell'Emilia-Romagna

da cui dipende anche Modena, è stata denunciata ieri anche dalla Garante regionale delle persone private della libertà personale, Desi Bruno. Sempre ieri, in una lettera arrivata all'ANSA, i detenuti del carcere di Modena hanno sottolineato le gravi conseguenze sulla loro vita quotidiana di questa situazione. Analoga lettera era stata inviata dagli internati della casa di reclusione di Castelfranco Emilia, nel settembre dell'anno scorso, al Ministero della giustizia. Sempre nel settembre 2015 i volontari della casa circondariale Sant'Anna e della casa di lavoro di Castelfranco Emilia spiegavano, in una lettera ai giornali, che tortura sia per i detenuti e gli internati di questi istituti penitenziari non riuscire a ottenere risposte dal magistrato di sorveglianza su temi importantissimi, come il permesso per un percorso di reinserimento (ad esempio, un lavoro all'esterno), per l'ingresso in una comunità o per un'alternativa alla detenzione; per non parlare del permesso di poche ore dopo anni di carcerazione, o il riconoscimento di quello sconto che la legge prevede e che permetterebbe di vedere ravvicinata la data del fine pena, oppure dell'autorizzazione ad uscire per fare volontariato o un lavoro di pubblica utilità, come - ancora una volta - la legge prevede. È proprio con le parole dei volontari, che faccio mie, che voglio concludere l'intervento. Quella del magistrato di sorveglianza è, per Modena, un problema inevaso da troppo tempo «per non lasciare un segno profondo nella credibilità delle istituzioni, quelle stesse istituzioni che hanno il compito di portare, attraverso la pena, le persone che con il loro reato si sono poste fuori dalla legge, ad averne rispetto e riporvi fiducia».